1.500/14, 1.500/15 e 1.500/16, in quanto tali proposte sono dirette a modificare il testo del disegno di legge

«a condizione che permangano i presupposti di cui all'articolo 1,». Si tratta, signor Presidente, della questione che riguarda l'attualità della pericolosità sociale, che è richiesta da tutte le sentenze della Corte di cassazione, secondo un'interpretazione conforme e uniforme, cui ha fatto riferimento lo stesso senatore Lumia nella sua replica.

delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo"». Credo che, per l'intelligenza da parte di tutti, abbiamo discusso in questi giorni che stiamo ragionando di un codice antimafia. Per cui noi siamo d'accordo, signor Presidente, che per tutti reati cosiddetti spia, che riguardano i reati contro la pubblica amministrazione, ove siano stati commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose, vadano correttamente applicate queste norme.

che correttamente a mio avviso avevamo richiamato nel precedente emendamento, del testo descrittivo per richiamare qual era la condotta che giustificasse quell'emendamento.

Non si è tenuto conto del fatto che esistono soggetti che hanno sì commesso un'evasione fiscale, ma che, in base alla legge, sono poi diventati legittimi possessori di quelle somme. Mi riferisco ai provvedimenti legislativi che riguardano lo scudo fiscale e altro. Domando: com'è possibile pensare che una somma che è diventata di legittima detenzione non possa essere impegnata.

kafkiana perché, da un lato, il Parlamento e la legge autorizzano la legittima utilizzabilità di quei soldi e, dall'altro, non ne teniamo conto. Alla fine, è evidente che il giudice arriverà a quella soluzione,

si tratta di misure cautelari che agirebbero in presenza di un avvio d'indagine anche per mere intenzioni delittuose, senza che queste abbiano una qualificazione riferibile al metodo mafioso o alla finalità di favorire un'organizzazione mafiosa. Non è difficile immaginare come queste misure cautelari possano essere ampiamente impiegate al di là della stessa finalità del legislatore.

si possa configurare un metodo mafioso nella commissione dei delitti indicati e che almeno uno di questi delitti sia effettivamente realizzato. Allo stesso tempo, altri subemendamenti sempre dedicati a circoscrivere la possibilità di applicare le misure cautelari

queste misure a carattere cautelare siano rivolte a persone per le quali non vi sia stato un giudicato definitivo, ma

posizione preconcetta o di schieramento, a valutare i profili di libertà che qui sono compresi

Quindi, perfino l'atto legislativo è stato considerato tra quelli configurabili nella qualificazione della corruzione.

di cui trattatasi, sia doverosa una cautela nel nome della libertà della persona, nel nome dell'*habeas corpus*, nel nome di diritti fondamentali che non possono essere conculcati solo perché il relativo provvedimento può dare

atti legislativi come fossero comunicati stampa, con finalità di mera comunicazione politica, laddove sono atti destinati poi a incidere sulla vita delle persone e delle loro famiglie.

poiché ho immaginato che i relatori, nello stendere il loro emendamento, il loro emendamento, si fossero sbagliati nel ritenere distinta l'ipotesi dell'articolo 640*‑bis* da quelle successive

già di per sé è un reato che va consumato in forma associativa. Ebbene, invito il sottosegretario Migliore, se ha un minuto di tempo, a inserire nel

che ha consumato il delitto in forma individuale. Vi faccio un esempio, perché uno l'ho scorto immediatamente: la truffa comunitaria. Il soggetto che, ai fini di ottenere un finanziamento dall'Europa, produce una serie di falsi documenti, sta operando da solo e la giurisprudenza lo vede condannato ai sensi dell'articolo 640*-bis*.

che mirano a realizzare una sorta di invalidità civili. Ebbene, quelle sono associazioni, ma il 640-*bis* può essere consumato anche in forma individuale. Sul punto,

Signor Presidente, io vorrei richiamare ancora una volta i colleghi al succo politico di questo provvedimento, illustrando il mio emendamento, 1.500/4. Esso prevede che per tutti i pubblici amministratori,

una legislazione speciale, che finora era riservata alle associazioni mafiose (e giustamente era eccezionale, era ai limiti o fuori della Costituzione, perché la piovra malavitosa in qualche modo andava, e va, colpita in maniera determinata),

poi vi sono trent'anni di tempo (primo grado, appello e Cassazione) che lo Stato prende per determinare se quel pubblico amministratore è o no colpevole degli addebiti che sono stati avanzati

mi sono limitato, per quanto si poteva fare, subemendando l'emendamento dei relatori, innanzitutto, come ha detto il collega Falanga, ad aggiungere agli altri reati per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Non si capisce, infatti, perché questo reato deve restare fuori dall'associazione, Oltretutto, è punito molto più blandamente di altri reati che invece richiedono l'associazione. In secondo luogo, mi sono permesso di togliere dall'elenco

di una erogazione, perché, se andate a vedere, sono reati puniti con pene da sei mesi a due anni. Cioè, rispetto ai reati di corruzione, sono fattispecie di cui, fra le altre cose, è facilissimo essere accusati. Come ho detto ieri, se non ci fosse il sindaco di Napoli, che è quello che è, se non vi fosse il presidente della Regione Puglia, che è quello che è, se non ci fosse il dottor Woodcock, che è quello che è, se non ci fosse una magistratura italiana, specialmente quella fatta

i pubblici amministratori se non i delinquenti che mettono già in conto di essere incriminati? Pensate che le persone perbene metteranno a rischio la loro vita, la loro famiglia, il loro patrimonio, il loro onore quando possono essere soggetti a misure di questo tipo?

perché estendendo a migliaia o a decine di migliaia di possibili fattispecie questa normativa speciale, evidentemente lo sforzo diretto dei tribunali e delle procure a combattere la mafia viene diluito e annacquato. Un conto è Totò Riina e un conto è è il peculato mediante profitto dell'errore. Noi li mettiamo sullo stesso piano? La nostra normativa diventa tutta speciale e va al di fuori delle regole dell'ordinamento? Spero almeno che questi emendamenti di riduzione del danno vengano accolti, fermo restando un giudizio finale che esprimeremo su una norma che comunque si pone sicuramente al di fuori delle regole costituzionali e soprattutto del buonsenso.

credo che il dibattito sia servito a molto, anche perché i relatori sono tornati sui loro passi e hanno preso spunto da alcune considerazioni che abbiamo fatto in Aula. Io non ci voglio credere, perché conosco bene i relatori avendoli ben frequentati in Commissione, ma mi sembra che l'emendamento 1.500 abbia fatto il gioco delle tre carte. Da una parte, cioè, si ha l'intenzione di rispondere sempre alla pancia del Paese, dall'altra parte ci sono le tirate di giacca della magistratura e dall'altra parte ancora

i relatori restringono la platea dei soggetti destinatari delle misure di prevenzione. Infatti, mentre il testo originario prevedeva che le misure di prevenzione fossero applicabili ai soggetti indiziati

(truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) e all'articolo 416 del codice penale, se finalizzati alla commissione dei reati previsti nella precedente versione. Pertanto, i reati contro la pubblica amministrazione

di prendere atto del buonsenso, però nella sostanza nella maggioranza vi è una posizione più morbida nell'applicazione delle misure di prevenzione per i reati contro la pubblica amministrazione, ma è come se tutto rientrasse dalla finestra.

a trovarsi, con delle situazioni che non possono essere sanate se non con un lungo periodo in cui il diritto viene sostanzialmente meno e la tutela

del complesso di queste misure, che andiamo a rivedere con il codice antimafia e che mirano soprattutto a scoraggiare, a limitare, a perseguire e infine a prevedere tutta una serie di delitti legati alla mafia, anche tutto quanto

si sono compiaciuti del fatto che all'interno di questo disegno di legge venissero ricomprese anche queste misure, proprio per bloccare, perseguire perseguire e mettere nel mirino una serie di comportamenti e di reati che sono estremamente dannosi per la salute del nostro Stato.

restringiamo. Elenchiamo una serie di articoli del codice per poi dire che tutti questi articoli del codice sono validi solo se passano attraverso un forellino piccolissimo.

Il rischio, con questa riscrittura, è che si faccia un passo indietro

il quale ha testualmente affermato, proprio con riferimento al testo del codice antimafia

dei delitti previsti dagli articoli 314 e seguenti in materia di pubblica amministrazione che, secondo l'attuale interpretazione giurisprudenziale, se caratterizzati dal requisito dell'abitualità, sono già compresi nella più ampia categoria di soggetti previsti dall'articolo 1, lettere *a)* e *b)*, del codice antimafia, articolo richiamato alla lettera *c)* dell'articolo 4.». Il procuratore nazionale antimafia Roberti «merita di essere segnalato il recente notevole incremento del ricorso alle misure di prevenzione personali e patrimoniali nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159. L'efficacia del sistema della prevenzione patrimoniale ha determinato una progressiva e crescente estensione della confisca a diverse tipologie di reati, se ed in quanto espressione di una abitualità a traffici illeciti ovvero produttivi di proventi tali da ritenere che i proposti i proposti vivano abitualmente con gli stessi». Ora, credo che se si vuole fare una lettura obiettiva

una specifica ipotesi legata ai reati contro la pubblica amministrazione quando questi fossero compiuti nel contesto di una truffa ai danni dello Stato o di una associazione

Onorevoli colleghi, è pervenuta alla Presidenza una richiesta di votazione a scrutinio segreto riferita ad alcuni subemendamenti all'emendamento 1.500, al voto degli articoli 1, 2, 5, 29 e 34, nonché al voto finale del provvedimento. Le richieste di voto segreto relative agli articoli 2, 5, 29 e 34 non sono ammissibili in quanto non ricomprese tra le fattispecie previste dall'articolo comma 4, del Regolamento. Inoltre, le richieste di votazione a scrutinio segreto su tali articoli sarebbero comunque risultate inammissibili a causa della loro tardività. Com'è noto, per prassi consolidata, le richieste di votazione a scrutinio segreto devono essere presentate in tempo utile affinché la Presidenza possa valutarle nel merito. Questo per ribadire il principio. La Presidenza ritiene invece ammissibili e tempestivamente presentate le richieste di voto segreto con riguardo agli emendamenti 1.500/2, 1.500/3,

1.500/11, 1.500/12 e 1.500/13, nonché all'articolo 1 nel suo complesso, in quanto tale disposizione estende l'ambito dei soggetti destinatari delle misure di prevenzione personali. Non è infine ammissibile, ai sensi dell'articolo 113, comma 7, del Regolamento, lo scrutinio segreto sul voto finale, in quanto le materie oggetto del disegno di legge risultano, per la maggior parte, al di fuori del novero di cui al precedente comma 4.

poc'anzi il senatore Pagliari, nel suo intervento, ha evidenziato che il procuratore nazionale antimafia ha mostrato la sua contrarietà all'allargamento della platea delle misure di prevenzione, ricordando come tutti i soggetti dediti a reati contro la pubblica amministrazione siano già destinatari di dette misure. Il relatore ha altresì affermato che il suo emendamento nasceva dalla constatazione che una cosa è commettere singolarmente il reato di corruzione e una cosa è, invece, commetterlo all'interno di un plesso associativo. Si può condividere o no questa impostazione, ma essa non può essere asistematica, cioè non può essere calata all'interno di un complesso dottrinario e giurisprudenziale che, per l'appunto, riguarda le misure di prevenzione.

si limita semplicemente a dire che quelle misure di prevenzione possono essere attivate nei confronti di chi è associato a un'associazione associato a un'associazione finalizzata al compimento di reati contro la pubblica amministrazione, a condizione

motivi sulla persistenza dei requisiti di cui all'articolo 1. Tutto qua, nient'altro che questo. In altri termini, si vuole rendere normativamente cogente per il giudice ciò che al momento è affermato solo dalla giurisprudenza, cioè sostanzialmente che per i reati diversi dall'associazione mafiosa e dai reati tipicamente mafiosi il giudice non deve muoversi per presunzione,

non capisco davvero la necessità di un parere contrario, a meno che la riserva mentale non sia quella di allargare alle misure di prevenzione per gli associati a le modalità indicate dalla giurisprudenza della Suprema corte per le procedure delle misure di prevenzione antimafia. Tutto qua. Davvero non riesco a comprendere la ragione del parere contrario. Pertanto invito i senatori, sia quelli che mi hanno ascoltato sia quelli che non mi hanno ascoltato, a votare favorevolmente sull'emendamento.

Intanto tutte le volte che si inserisce, quanto all'applicazione delle misure di prevenzione, non soltanto il riferimento all'articolo 416-*bis*, ma anche il riferimento all'aggravante di cui all'articolo 7 sostanzialmente non si introduce alcuna innovazione, perché l'articolo 416-*bis* sta all'interno dell'articolo 4, cioè è una disposizione la quale rende già immediatamente applicabili le misure di prevenzione. Analogamente si deve dire per l'articolo 7, ossia l'aggravante della finalità di agevolare le organizzazioni mafiose, ovvero dell'avere agito con metodo mafioso, in quanto è contenuto nell'articolo 51, comma 3-*bis* del codice di procedura penale richiamato dall'articolo 4. Quindi tutte le disposizioni che introducono il riferimento o all'associazione di stampo mafioso ovvero all'aggravante in realtà non fanno altro che replicare quanto già oggi esiste, quindi non sono dotate di capacità modificativa del testo in quanto già oggi, in presenza di questi presupposti, le misure di prevenzione sono applicabili.

prego le colleghe e i colleghi di riflettere in coscienza su questo emendamento e su quelli che seguiranno perché hanno l'obiettivo essenziale di circoscrivere misure significative come quelle rivolte a limitare la libertà della persona e il suo diritto di proprietà in relazione a una mera fase indiziaria. Qui si propone di sostituire il termine «indiziati» con il termine «imputati» affinché vi sia

Il senatore Sacconi dice che si devono attivare le misure di prevenzione nei confronti degli imputati e non nei confronti degli indiziati, così come invece accade secondo questa disposizione. Ma la realtà di fondo, signori, è che la categoria degli indiziati è una categoria diversa rispetto a quella degli indagati e a quella degli imputati. E allora chiariamo chi sono. L'indagato è un soggetto nei cui confronti ci sono degli elementi per iscriverlo al registro notizie di reato e promuovere nei suoi confronti un'indagine. L'imputato è una persona nei cui confronti viene esercitata l'azione penale, che quindi sostanzialmente avrà un suo sfogo dibattimentale. L'indiziato non è un indagato e non è un soggetto nei cui confronti si sia aperto un procedimento penale, ma è un'altra cosa. Il che evidentemente credo - e ringrazio il senatore Sacconi per questo emendamento - disvela una grande verità: queste misure di prevenzione si muovono nei confronti di un sospettato. Quanto poi questa azione possa essere sintonica con uno Stato di diritto, come almeno a parole continuiamo ad affermare di essere, questo non è chiaro.

credo che vada ricordato come l'impostazione del sistema delle misure di prevenzione abbia ormai superato il vaglio della Corte di cassazione, della Corte costituzionale e di tutte le corti europee, perché viene impostato proprio sulla necessità di una tutela avanzata e di una tutela preventiva nei confronti di reati particolarmente gravi. Relativamente a questi reati particolarmente gravi di mafia, di grande criminalità organizzata, di terrorismo e alcune tipologie che sono indicate, è già stata ammessa la possibilità di questa sorta di cosiddetto doppio binario, a tutela della società, a tutela della sicurezza dei cittadini e della nostra collettività. Quindi questa proposta di rispostare in avanti la tipologia dei reati per i quali siano ammesse le misure di prevenzione è assolutamente da non accettare, proprio per quello che è lo stato della nostra legislazione antimafia antiterrorismo e per quella che è la giurisprudenza ordinaria e costituzionale.

per sottolinearlo con forza e per invitare anche gli altri a sottoscriverlo, sia per il discorso che è stato fatto sullo Stato di diritto, sia perché mi viene anche un po' da sorridere, perché poi quando le incertezze le incertezze prendono il sopravvento si vedono le cose diversamente. La giustizia è una ruota che gira, signori miei; quindi certi impulsi giustizialisti, che poi spesso si ritorcono contro nel tempo e provocano una revisione delle cose, aggravano anche la confusione e la sfiducia dei cittadini. Quindi sottoscrivo convintamente questo emendamento. Presidente, credo che l'Assemblea stia affrontando questi problemi con una leggerezza fuori dal comune. Infatti si continua tranquillamente a parlare, perché in Italia pensiamo a ben altro e non ai veri problemi che attanagliano questo Paese, e uno di questi problemi è la giustizia. E li affrontiamo nella maniera più sbagliata,

E per questo gli viene confiscato tutto? A quanta gente è accaduto? A quanti amministratori? Io certamente d'ora in poi non consiglierò a nessun mio amico di fare il consigliere comunale o altro, perché lo mando incontro forse alla fine della sua vita.

perché al delinquente incallito sapeste quanto gliene importa poco di quanto stiamo facendo. Come diceva qualcuno, meglio mille ladri fuori che un solo innocente dentro. Questa massima non vi appartiene. Siamo fuori: lavoriamo per i cittadini o per le fisime?

chi sta da una parte non istituzionale ma di un ordine che vuole sempre di più. Non credo che la politica e i rappresentanti dei cittadini debbano delegare ad altri il futuro e la serena vita di cittadini che fanno il loro dovere. Riflettete bene.

dicendo che per la mafia non era necessario un elemento di accertamento. Per il terrorismo avevamo usato un'espressione - che poi ci è stata confermata in Commissione coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero

cui si dice che tizio è indiziato di uno dei reati verso la pubblica amministrazione ed è indiziato anche per il 416?

Volete farmi credere che questo risponde a principi di civiltà giuridica? Leggete quanto hanno scritto sulla questione i professori universitari e gli interpreti del diritto in questo fine settimana. Signor Presidente, Signor Presidente, proprio per la sua storia, avevo presentato un emendamento - ce ne sarà un altro subito dopo - per riscrivere questo testo. Un conto è dire che quelli sono i reati spia della mafia, per cui dobbiamo combatterla dobbiamo far sì che quei reati siano colpiti quando vengono posti in essere per agevolare le associazioni mafiose. Ma, quando si tratta di un cittadino comune e di un reato comune, che cosa risolviamo? Con parole come «indiziati» abbiamo un embrione di uno stato di polizia contrario a quelle che sono le regole della nostra democrazia, contrario a quelle che sono le regole del processo penale.

parte di questa Assemblea nella passata legislatura - quando per cinque mesi scrissi questo codice insieme ad altri. E questo codice doveva servire a combattere la mafia.

Senatore Caliendo, è inutile che lei richiami la mia precedente funzione perché adesso è un'altra. Non posso esprimermi nel merito,

perché nel processo di prevenzione non esiste uno *standard* probatorio e, quindi, il legislatore si esprime con un termine intermedio che, per l'appunto, è il termine indiziato, che è sempre esistito. Quanto poi alla distinzione tra indagato e imputato, è una distinzione fondamentale - non credo di dover intervenire - perché riguarda soltanto la fase processuale: si diventa imputati quando c'è un rinvio a giudizio pronunciato dal giudice. Mi permetto, però, di intervenire ulteriormente. Il sistema delle misure di prevenzione si regge sostanzialmente su un doppio canale di accesso. Sul versante dell'articolo 1, si può essere sottoposti a misure di prevenzione se si è dediti a delitti, ovvero se si viva, anche soltanto in parte, dei proventi di attività illecite. Trascuro ovviamente il successivo articolo 3, perché poco rilevante su questo versante. In sostanza, le misure di prevenzione, per quanto riguarda l'articolo 1, implicano attività reiterate. poi l'articolo 4, che riguarda un sistema per cataloghi di reati. L'articolo 4, cioè, che è collegato all'articolo 1, anche in virtù dell'articolo 16, al contrario, prevede singoli reati. Storico è l'articolo 416*-bis*, ma ovviamente sul punto nessuno può esprimere alcuna osservazione. Devo poi notare che nel 2008 e nel 2009, con i pacchetti sicurezza, si è dilatata la categoria numerica dei reati che singolarmente possono comportare l'applicazione delle misure di prevenzione, introducendo il tifo violento e la ricostituzione del partito fascista. il cosiddetto codice antimafia non sia poi del tutto un codice antimafia nasce già nel 2008-2009 ed è poi reiterato con la versione definitiva del 2011. di osservazioni e di riserve di natura sistematica per quanto riguarda la dilatazione per categorie di singoli reati del cosiddetto sistema antimafia, del codice antimafia. non si distinguono le misure di prevenzione dalle misure di sicurezza, perché è difficile il giudizio di pericolosità sociale e quant'altro. Il punto giuridico, ma anche politico, di questa mia affermazione è che l'emendamento presentato dai relatori si giustifica proprio su questo versante. Proprio per non aver voluto accedere a un codice antimafia per titoli di reato, per come era nella soluzione consegnataci dalla Camera, i relatori hanno presentato un emendamento il quale, al contrario, lega la misura di prevenzione a un contesto organizzato di tipo criminale, ancorché non di tipo mafioso. Ma quello non lo si poteva fare e io l'ho già detto poco prima perché, se lo si fosse fatto, si sarebbe introdotta una norma esistente, e ovviamente non si poteva fare. Immagino che nelle scelte fatte dai relatori si sia dovuto individuare quel contesto associativo non di stampo mafioso, e che quindi introduce una disposizione innovativa, che lega i delitti contro la pubblica amministrazione a un contesto associativo. È chiaro che chiaro che poi il Senato si regolerà nelle sua massima libertà morale nello scegliere l'una versione o l'altra. Il contesto associativo, intanto, introduce una componente temporale tipica di un sistema che impone la reiterazione delle condotte. L'articolo 416 del codice penale prevede un reato per l'appunto permanente, dove la componente cronologica temporale la fa da padrona. Quindi, in un certo senso, è un sistema assonante sia con l'articolo 4 nella parte in cui richiama l'articolo 416-*bis*,

un programma indeterminato di delinquenza, significa agire proprio nella direzione della prevenzione, ossia della interdizione di una struttura associativa funzionale alla commissione di un numero indeterminato di delitti che, se interdetta, non commetterà più Questo per dire che l'emendamento presentato dai relatori è conforme allo spirito del codice antimafia. Non lo sarebbe stato se fosse stato un sistema per singoli titoli di reato, per come i relatori hanno ritenuto di dover impedire che fosse, perché in quel caso si pongono problemi di sovrapposizione tra misure di prevenzione e misure di sicurezza, che è un grosso problema giuridico, e soprattutto quella difficoltà di selezionare il concetto di pericolosità sociale che, sulla base della commissione di un unico reato, ovviamente sarebbe stato difficile individuare. Ciò, però, non è per le fattispecie associative, le quali sono la concretizzazione proprio dell'idea del pericolo. Per queste ragioni mi permetto di esprimere una parola a sostegno dell'emendamento presentato dai relatori.

Confermo, quindi, una progressiva dilatazione di una strumentazione eccezionale, nata per combattere la mafia

il senatore Casson, che se ne intende - si pone però all'interno di una logica di difesa avanzata. Per cui, come nell'Unione Sovietica per i reati contro il socialismo si poteva finire in galera, perché sospettati di voler colpire le istituzioni; o come, durante il fascismo, c'erano le leggi speciali, qui si introduce il concetto che un cittadino amministratore

ex deputata e ricercatrice, travolta da accuse infamanti riguardanti la pubblica amministrazione, accusata di aver lucrato o di voler lucrare non so quanti miliardi sulla pelle della salute degli italiani e fatta oggetto di una campagna scandalistica de «L'Espresso»?

capire che le misure eccezionali che riguardano la mafia, la 'ndrangheta e la camorra non possono essere applicate sulla base di un sospetto? Come ripetutamente leggiamo nelle informative di polizia: non si può escludere

Mi sembra che ne ce ne sia abbastanza per una riflessione su un chiarimento. E, se si decide di scrivere la parola «imputato», si rientra nel novero dei Paesi civili dell'Occidente; ci si allontana dal comunismo, dal fascismo, dalle leggi speciali e si rientra nell'ambito di un concetto di giustizia per il quale anche la pena più severa (patrimoniale o meno, detentiva o meno) viene applicata a una persona riconosciuta colpevole di aver commesso un reato e non soltanto sospettato, in una posizione difficile come quella dei pubblici amministratori. Andate a vedere le vicende che hanno coinvolto amministratori di tutti i partiti, da Sesto San Giovani a Roma, al Sud,

facciamo qualcosa che già in maniera pregiudiziale ha distrutto una persona, a prescindere dal fatto se poi verrà riconosciuta colpevole o innocente. Volete che il Parlamento italiano voti una disposizione del genere?

che abbia commesso qualcosa che non andava. Certo, se i casi come quello della nostra collega Capua non insegnano niente, c'è veramente da essere disperati sul futuro del nostro Paese. pochi minuti fa ho suggerito al sottosegretario Migliore e al relatore Lumia di andare a controllare il

Non hanno voluto farlo e hanno bocciato il mio emendamento. E, quindi, mi sono permesso di far stampare solo due sentenze - ma ce ne sono migliaia nel repertorio della Cassazione italiana - dove c'è la condanna ai sensi sensi dell'articolo 640-*bis* di un solo soggetto. Non avete neanche l'umiltà di andare a controllare, non fosse altro per la funzione istituzionale che ricoprite. Avete l'obbligo di studiare perché, se non lo fate e restate ignoranti, danneggiate il nostro Paese e gli italiani.

senza che questo in alcun modo voglia rischiare di rasentare il voto di scambio, vorrei proporre un accordo ai

per ancorare le misure di prevenzione a un reato associativo di carattere permanente che, in quanto tale, manifesta la sua pericolosità. Non comprendo - devo dire la verità - la prima questione: se il problema è il reato associativo, perché le misure di prevenzione antimafia si applicano ai reati contro la pubblica amministrazione e non vengono associazioni a delinquere per rapine, estorsioni e tanti altri reati gravissimi forieri di profitti criminali? Ho quindi l'impressione che l'aspetto associativo

il senatore Caliendo, citando un collega - che, se tutto è mafia, nulla è mafia. Il problema - secondo me - non è neanche questo. Il problema è che, se noi utilizziamo gli strumenti non ordinari per il contrasto alla criminalità mafiosa per tante altre forme di criminalità, andiamo a indebolire il contrasto alla criminalità mafiosa Ciascuno di noi sa quanto tempo occorre per svolgere in maniera corretta gli accertamenti patrimoniali e bancari, che sono il presupposto per la misura patrimoniale antimafia. E tutti quanti noi sappiamo come purtroppo spesso le Forze dell'ordine impegnate nel settore, con la loro specificità, patiscono dei ritardi nelle risposte proprio in ragione della massa di lavoro rispetto alla quantità di energie investigative. Non vi rendete conto che dare la possibilità di attivare una misura di prevenzione antimafia nei confronti di criminali - senz'altro - che però con la criminalità mafiosa nulla c'entrano, significa consentire a qualsiasi ufficio giudiziario d'Italia di impegnare le Forze dell'ordine - penso in particolare alla Guardia di finanza - in attività che forse potrebbero essere con maggior profitto spese nel contrasto alla criminalità organizzata. Ho sentito discussioni su indiziato e indagato e sulle leggi del 1965 e del 1982. Nel nostro codice, però, noi abbiamo - come dicevo prima - l'indagato e l'imputato; l'indiziato è una categoria a parte. Sicché si potrebbe verificare la seguente situazione: un soggetto iscritto a registro notizia di reato, e quindi indagato per il reato di corruzione, indiziato in ragione di una denuncia della polizia giudiziaria per associazione a delinquere, può essere sottoposto a misura di prevenzione anche se non ha mai subito un procedimento per il reato di associazione a delinquere, essendo pacifico che è indiziato per lo stesso.

al di fuori dell'obiettivo che deve essere focalizzato, significa in qualche modo indebolire la lotta alla mafia. Ed è per questo che abbiamo proposto l'emendamento

che hanno commesso reati contro la pubblica amministrazione, in quanto spesso sono reati spia, e cioè sostanzialmente segnalano la vicinanza tra l'amministratore pubblico e la criminalità organizzata mafiosa. Apro e chiudo una parentesi: senatore Zanda, se c'è un reato spia, è esattamente quello che voi - a mio avviso, forse giustamente - a tutela dei sindaci non avete inserito, ed è l'abuso in atti d'ufficio patrimoniale. Il vero reato spia è esattamente quello che stranamente non vedo tra quelli previsti.

e cioè se vengono posti in essere secondo le modalità di cui all'articolo 416-*bis*, ovvero se sono finalizzati alla vita di quella associazione. Nient'altro che questo. Io credo che, nel votare a favore di questo emendamento, noi faremmo un grande favore al contrasto alla criminalità organizzata in quanto, puntando - sì - sui reati contro la pubblica amministrazione, ma qualificati dalla loro correlazione con la criminalità organizzata, spenderemmo bene le energie investigative a disposizione. lei ha precedentemente detto che questo è un provvedimento strategico per il Partito Democratico. Immaginavo che fosse così. Noto che è un provvedimento strategico per la maggioranza,

si fa riferimento al metodo mafioso con cui si dovrebbe realizzare il processo criminoso che viene ipotizzato,

a ipotesi di reati contro le cose che non hanno quella qualificazione straordinaria che può legittimare misure altrettanto straordinarie. Prego le colleghe e i colleghi di riflettere davvero su ciò che stiamo decidendo per il futuro della nostra società.

in questo caso l'emendamento ha una modesta, ma ancora significativa portata, ossia quella di richiedere che, per

i diritti dei cittadini a qualcosa che abbiano commesso di reale e penalmente rilevante, vengono cancellati sulla base dell'antica teoria che il diritto del singolo, anche se innocente, va sacrificato Ce l'hanno già raccontato il nazismo, il fascismo, il comunismo e oggi ce la raccontate di nuovo.

perché voi state ritoccando le minime garanzie di uno Stato democratico. Se si tratta di fare la lotta alla mafia e alle organizzazioni criminali, Forza Italia

Con l'emendamento 1.500/13 voglio fare un ultimo tentativo per rendere funzionale e coerente con il sistema l'emendamento dei relatori. Non lo modifico,

perché, se così non è, aprite un varco enorme. Nessuno farà più politica. Nessuno avrà più il coraggio di candidarsi alle elezioni amministrative nel nostro Paese. Già così trovate difficoltà. Non devo nemmeno dirvi di stare attenti, perché questo è un altro argomento di campagna elettorale e perché voi state attentando ai diritti dei cittadini e alle garanzie previste dalla nostra Costituzione. Qui mantengo in piedi l'emendamento dei relatori. Non ne chiedo la modifica. Vi chiedo di aggiungere che quei reati

favore, perché avremo la necessità di garantire comunque un intervento. Allora, se avete una coscienza, nel voto segreto ragionate sulla possibilità

quando avrete realizzato un'operazione di questo tipo. L'aggravante serve soltanto a dare un ulteriore, forte potere alla Direzione nazionale antimafia

il Movimento 5 Stelle è contrario all'emendamento 1.500, perché la previsione del reato associativo restringe di molto l'ambito di applicazione della norma, così come è stata approvata in Commissione. Il fenomeno corruttivo è un'emergenza nazionale ed è inutile che lo ribadisca, ma lo è non per colpa del Movimento 5 Stelle. È giusto intervenire con priorità e il provvedimento in esame va in quella direzione, soprattutto l'articolo 1. dei relatori, però, è troppo restrittivo, rispetto - ad esempio - ai responsabili di singole e gravi condotte di appropriazioni di soldi pubblici. Inoltre, renderà molto difficile provare l'associazione finalizzata, come - ad esempio - il peculato.

la previsione approvata dalla Commissione, essendo più ampia, è sicuramente più rispondente

Camera. Ritengo sia preferibile il testo così come uscito dalla Commissione. Mi domando come mai il Movimento 5 Stelle, che

una maggiore ampiezza. Così come è curioso che l'emendamento che riportava una maggiore ampiezza sia stato votato favorevolmente da Forza Italia, che immagino accetterà altrettanto questa restrizione che l'emendamento dei relatori implica. Io credo che tutti questi giochetti non facciano bene alla lotta contro la mafia.

perché considero l'emendamento dei relatori sostanzialmente ininfluente dal punto di vista della limitazione delle libertà che con questo provvedimento si produrrà. Penso davvero che non abbiano luogo le preoccupazioni che ho sentito esprimere dalla collega del Gruppo Misto. Non sfuggirà la notevole discrezionalità con la quale con la quale possono essere definiti gli indizi in base ai quali un soggetto verrà imputato imputato di mere intenzioni che vorrebbe realizzare attraverso un'associazione a delinquere per la quale non serviranno molti argomenti, ma solo labilissime indicazioni.

Questo è indubbiamente un emendamento, quindi credo che si debba fare il procedimento corretto per un emendamento. Oltre tutto, se non si parlano prima il Governo e i relatori, non è colpa dell'opposizione. Senatore Volpi, la Presidenza è rimasta assolutamente sorpresa dal fatto che tra relatori e Governo non ci sia questa

la valutazione della proposta di riformulazione è un'altra questione.

No, semplicemente noi sapevamo che avrebbe fatto questa proposta di riformulazione del «Conseguentemente (...)» e quindi il senatore

Non so se sono stato chiaro. Se è un nuovo emendamento, c'è la facoltà di subemendare; se è una riformulazione, si può accettare, ma è una valutazione della Presidenza.

Presidente, la storia repubblicana era abituata in quanto a giustizia a un altro Migliore. Questo non mi sembra si possa paragonare con il Migliore.

Non è possibile. Se c'è un problema che riguarda i banchi del Governo, interrompa la seduta. Non può dare suggerimenti nel senso che domanda al Sottosegretario se ci sono altri emendamenti e il rappresentante del Governo si gira e le dice una cosa che non sentiamo. Interrompa la seduta.

Per quanto riguarda la mia disattenzione, non mi pare; anzi, c'è un eccesso di attenzione.

c'è stata una proposta diretta del Governo di un emendamento. Si tratta di emendamenti: che non si facciano le furbate di far proporre in modo diverso le stesse cose, perché questa Assemblea si sentirebbe presa in giro.

c'è stata una proposta, sempre da parte dello stesso rappresentante del Governo, di modificare o introdurre - non ho capito bene - un comma 3, un comma 4. Ripeto, non ho capito se questa è la proposta del Governo o se è un invito

Le altre cose sono aggiuntive, sono qualcosa in più che non capisco perché vengano proposte. A questo punto vorrei capire se il Governo fa una proposta di riformulazione,

attribuisca questo potere alla Presidenza, indubbiamente, ma su espressa richiesta del Governo o della Commissione.

Nell'interesse della discussione, il Presidente può decidere l'accantonamento e il rinvio. Quindi, il Presidente può decidere l'accantonamento ma sospendendo la seduta e rimandando il provvedimento eventualmente in Commissione. Mi pare

Presidente, l'emendamento dei relatori 2.300 si conclude con: «Conseguentemente, all'articolo 12 sopprimere il comma 2*».* Domando a lei, che ha ammesso l'emendamento: a quale comma 2 si riferisce?

non ha nulla a che fare con la norma appena introdotta dall'emendamento. Potrebbe avere qualcosa a che fare con il comma 3, se il secondo

e lo può fare, l'accantonamento di tutto l'articolo 2. Quando sarà chiaro che cosa vogliamo eventualmente riformulare o modificare, allora potremo avere la chiarezza per andare avanti e decidere di conseguenza.

tratta una questione che i relatori conoscono benissimo. Mi aspettavo un parere favorevole dei relatori e del Governo su di esso.

per quanto riguarda le misure di prevenzione antimafia, vi è una competenza propria del procuratore distrettuale, del procuratore anche del luogo della dimora e, volutamente, come lei ricorda meglio di me,

Questa è la soluzione più corretta, perché, altrimenti, si grava il procuratore distrettuale antimafia di una serie di compiti che, invece, vengono svolti dal procuratore circondariale. del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sono attribuite al procuratore della Repubblica presso il tribunale del circondario, previo coordinamento con il procuratore della Repubblica distrettuale. Perché?

che se tutti e due potevano svolgere la stessa funzione si sarebbe aggravato il lavoro di entrambi, perché l'uno non sapeva quello che faceva l'altro. l'attuale sistema garantiva al procuratore distrettuale una maggiore attenzione e libertà di movimento sulla mafia, lasciando al procuratore circondariale questa attività.

altresì verificato che anche la votazione dell'articolo 3 è connessa all'articolo 2, annullo la votazione dell'articolo 3.

Presidente, io prima volevo chiedere, ma non mi sono permesso, se eravamo certi che le votazioni che stavamo facendo non avessero una connessione. Mi permetto di dire

si interpreta questa nostra proposta come un nuovo emendamento, ritiro la proposta di riformulazione ed esprimo parere favorevole

che anche all'Assemblea interessi, ma interessi votare un certo testo. Abbiamo fatto una serie di votazioni successive all'accantonamento, di cui adesso dobbiamo disporre la cancellazione. Io non credo sia una buona cosa varare le leggi votando degli articoli e cancellandone l'approvazione perché era subordinata all'approvazione dell'articolo 2.

detenuti, ma anche gli ammalati e l'impossibilità di essere presenti, perché sopprimiamo anche l'ultimo aspetto che viene ancora preso in considerazione? Non riesco a raccapezzarmi e mi sembra che sia inutile sopprimere.

Signor Presidente, poi vedremo con il Gruppo come votare su questo emendamento, ma una cosa sinceramente non riesco a comprendere. Il Governo presenta un emendamento, quindi io immagino

una correzione. Come può politicamente sostenere che lei ritira l'emendamento perché era considerato un emendamento e quindi non serve più? O serve oppure non serve. Guardi che politicamente non è che sta facendo una bella figura.

si metta un po' d'accordo con se stesso; non mi riferisco a lei personalmente, ma al Governo. Se il Governo presenta un emendamento e poi lo ritira con queste motivazioni, credo che sia un fatto estremamente grave. E lo dico anche ai colleghi della maggioranza. ci spieghi, ci faccia il favore di spiegarci cosa voleva fare prima e perché adesso non vale più. Solo perché non potevamo fermarci per portarlo in Commissione bilancio

Il problema poi è la valutazione nel merito, che spetta alla Presidenza. Adesso il Governo ha ritenuto di ritirarla. Io apprezzo la sua valutazione dal punto di vista politico, senatore Volpi, però la sua rimane una valutazione.

individuando come destinatario della norma soltanto il direttore di cancelleria, ovvero ha modificato la platea dei destinatari della norma. A me non pare che possa trattarsi di una riformulazione. Si va a ridurre il numero dei soggetti

Presidente, vorrei ricordarle che il Regolamento e la relativa prassi introdotta al Senato prevedono che prima degli emendamenti ad ogni articolo venga richiamato il presentatore. Questo serve per Questo serve per richiamare anche l'attenzione dei senatori presenti sui presentatori dei vari emendamenti e dei relativi Gruppi di appartenenza. Mi sembra che non seguire questa prassi introduca una maggiore confusione, anche se sono d'accordo che forse quel continuo richiamo

dove si procede con grandissima generosità a sequestri, a blocchi, questo emendamento, nella sua stessa formulazione, ricorda che non sono cose indolore. Non è che più si sequestra,

nelle sue origini legittime, dal fatto di rendere giustizia ai cittadini e non dal fatto di esercitare il potere nei confronti dei cittadini - sono due concezioni diverse dello Stato su cui temo che ancora non ci sia

sale a livello più basso di tutta l'Europa. Strano, davvero strano. Si minacciano tutte le attività economiche in ogni modo: si pensi ai reati

ha rilevato che vi sono, in particolare in alcune zone (ma in realtà dappertutto),

Il problema c'è: sequestra, sequestra, sequestra e poi, stranamente, in certe zone l'unico datore di lavoro magari è la mafia. Per forza: tutte le altre attività vengono bloccate. E poi si trova strano il fatto che la mafia riesca ancora a reclutare qualcuno, nonostante i colpi, pesantissimi, che meritoriamente sono stati dati a queste organizzazioni criminali.

Vorrei infatti sapere quale territorio del nostro Paese non presenti particolari fragilità economiche e sociali. E noi lo aiutiamo rendendo possibile il sequestro e il blocco dei beni e rovinando le persone. per qualcuno questo può essere solo un gravissimo disagio, per un imprenditore il blocco dei beni, il sequestro, l'obbligo di risiedere in una certa località o di non risiedere in una certa località significa distruggere la sua azienda. Qualcuno si è il posto il problema, e rendo merito alla collega che ha presentato l'emendamento. Altri, evidentemente, questo problema non se lo pongono, perché non importa se si aumenta la disoccupazione; non importa se si deviano ulteriori investimenti in altri Paesi; non importa se si scoraggiano gli investimenti. L'importante è dare

infatti, di dover insegnare a nessuno che gli uffici giudiziari hanno necessità di indipendenza e imparzialità, che riguardano non solo i magistrati

intende escludere il personale di cancelleria dalle persone che possono essere tali da condizionare quel procedimento attraverso propri creditori, debitori, eccetera.

Tuttavia togliere il personale di cancelleria significa né più né meno che tutte queste operazioni, come è avvenuto in qualche caso, possono essere realizzate attraverso il personale di segreteria addetto al magistrato. Signor

magistrato, ma anche il personale di cancelleria. Se vogliamo inserire il dirigente e il presidente del tribunale sono d'accordo, ancorché non svolgano attività diretta. Altrimenti,

una resipiscenza da parte dei relatori e non perché vogliamo fare ostruzionismo. Vi rendete conto che scrivere la parola: «dirigente» non ha senso rispetto all'obiettivo che vogliamo raggiungere?

significa limitare a forse un caso di dirigente che assiste il magistrato. La dicitura: «personale di cancelleria che assiste», indipendentemente dalla qualifica, comprende sia il dirigente sia il personale che normalmente assiste Signor Presidente, l'idea di proporre l'emendamento 13.104 è venuta all'esito di una discussione che abbiamo avuto in Commissione giustizia quando abbiamo analizzato i tantissimi risvolti del provvedimento che sono stati oggetto di confronto e di discussione. Ricordo che in tema di incompatibilità degli amministratori giudiziari e dei rapporti che tra questi intercorrono, o possono intercorrere, con i magistrati affidanti si era sviluppato un dibattito e io avevo anche proposto - non so se lo si ricorda - l'adozione di un sistema di incompatibilità pari a pari a quello dell'astensione obbligatoria previsto dall'articolo 51 del codice di procedura civile, che era il senso dell'emendamento che ho ritirato. Il ritiro dell'emendamento

in seguito ad una serie di discussioni con delle organizzazione sindacali in Sicilia, che lamentavano la rovina cui spesso andavano incontro le aziende che venivano confiscate, con le conseguenze che possiamo immaginare sul personale che in quelle aziende lavorava.

l'Agenzia, entro un mese dalla comunicazione della confisca definitiva, pubblichi sul proprio sito Internet l'elenco dei beni immobili oggetto di confisca. Nell'emendamento si propone di aggiungere, oltre a quello dei beni immobili, anche l'elenco delle aziende confiscate con l'indicazione analitica ed estimativa delle attività e della situazione patrimoniale, economica, finanziaria e produttiva.

esiste anche il problema, per quanto riguarda le aziende, che la gestione, per come è stata condotta in questi anni, assegnata spesso ad un amministratore giudiziario unico per più aziende, quindi è una gestione obiettivamente fatta male,

a determinare la rovina di queste aziende, con il licenziamento del personale, la perdita di posti di lavoro e tutto il resto. Si tenga conto che su questo tema ho già presentato in più occasioni delle segnalazioni al Governo,

tanto che si venivano a creare delle condizioni per cui delle aziende funzionanti, efficienti e produttive

Se noi riuscissimo ad avere la possibilità di una valutazione precisa del bene che va ad essere confiscato, diventerebbe più semplice individuare le responsabilità di chi lo ha fatto deperire.

proporre ai colleghi una colletta in favore del senatore Pagnoncelli che non è presente in Aula e ha dovuto lasciare una pallina di carta a votare al suo posto. Il furbetto del cartellino di oggi

Meglio ancora, concerne il fatto che abbiamo una situazione di grave pericolo di inquinamento di una perla della nostra struttura ambientale. Per le operazioni di ripristino, infatti, sono stati utilizzati dei sacchi di cemento Abbiamo presentato un'interrogazione un anno fa su queste problematiche. A distanza di un anno le uniche notizie che abbiamo è che queste tonnellate e tonnellate di polvere di cemento si stanno depositando sui fondali danneggiandoli in maniera irreparabile e gli esperti dicono che non sarà possibile

in termini di occupazione e di mancata restituzione del prestito sociale. È un problema di grandi dimensioni che impone sia misure che risposte urgenti ma anche risposte di indirizzo che il Governo deve dare per rivedere i nuovi strumenti di controllo affinché non capiti più che vi siano risparmi di intere famiglie che non vengono restituiti. Serve una riflessione. Chiedo che questa interpellanza, che è stata depositata il 16 maggio scorso, venga calendarizzata in Aula al più presto. **Sulla mancata

fino quando non avrò una risposta chiara. Voglio sollecitare a procedere velocemente alla nomina dei senatori che devono comporre la Commissione monocamerale d'inchiesta sulla ricostruzione postsisma dell'Aquila.

il quale sarebbe stato molto importante per fare un lavoro incisivo, oltre che per chiarire alcune vicende poco trasparenti legate alla ricostruzione e all'utilizzo dei fondi stanziati. La collega Montevecchi, che allora ricopriva la carica di Capogruppo, su richiesta, indicò il mio nome e quello del senatore Castaldi come componenti della Commissione d'inchiesta Nulla si è ancora saputo dei nominativi indicati dagli altri Gruppi. Non si sa se tutti abbiano dato le loro indicazioni e se alcuni ancora non hanno trasmesso l'indicazione dei nominativi forse per meri calcoli elettoralistici, legati legati alla tornata di elezioni amministrative appena passata. Speriamo che adesso si sentano più liberi - ovviamente la mia è un'ironia - e procedano a dare le loro indicazioni. Questa dilazione dei tempi è molto difficile da giustificare e motivare con ragioni diverse da una totale assenza di volontà politica. Con il mio intervento, pertanto, le chiedo, signor Presidente, ai sensi dell'articolo 2, del documento che istituisce la Commissione d'inchiesta, di procedere il prima possibile alla nomina dei componenti, sollecitando i Gruppi parlamentari a proporre i senatori che intendono far parte della Commissione o, in alternativa, di indicare le ragioni o i Gruppi parlamentari che finora hanno di fatto impedito l'avvio di questa importante Commissione d'inchiesta. Avviarne rapidamente i lavori era ed è un atto doveroso verso i cittadini aquilani e la legalità.